necessitavo di cinque minuti; oggi sarebbero sufficienti trenta secondi, oppure ci vorrebbe una buona mezz'ora, per affrontare quello che è successo. Partiamo dal metodo. Ieri, ad un certo punto, dopo le relazioni di maggioranza e di minoranza è stato presentato un maxiemendamento, così lo definirei, da parte del Governo su un provvedimento che si intitola «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2006 n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo». Il maxiemendamento di tutto parla tranne che di questo; il presidente Schifani, invece, ha detto che, siccome si trattava di questioni relative ai trasporti, la materia era in qualche modo relativa a questo tipo di discorso. Benissimo, c'è una decisione politica presa dalla gestione della nostra Camera,

privati piuttosto che con il servizio pubblico, che deve garantire i trasporti e che era al centro di buona parte del decreto‑legge che oggi ci troviamo Dico privati perché è difficile in Italia inquadrare in questa categoria qualsiasi tipo di imprenditoria, visto e considerato che da una parte si disegnano misure che in qualche modo tolgono qualsiasi rischio d'impresa, fissando sempre, solo e comunque quote minime e andando ad aiutare qualsiasi tipo di categoria e, dall'altra, si cerca sempre di infilare comunque una componente politica ogni qualvolta si ha a che fare con questioni attinenti al mercato del lavoro ed alla libera concorrenza. Questo Governo, che ha la parola libertà nel nome della parte politica fondamentale che lo sostiene in Parlamento, ad oggi, non è riuscito a proiettare un minimo di idea su che cosa si intenda fare in materia di liberalizzazioni, di libero commercio, di libera concorrenza e anche di libera contrattazione. Non mi soffermerò sul maxiemendamento, perché so che i colleghi del Gruppo del PD vi hanno molto lavorato. Va anche ricordato che sono state date sei-sette ore scarse per elaborare

Mi soffermerò invece sulla questione Tirrenia, utilizzando buona parte di un articolo pubblicato qualche settimana fa dal segretario dei Radicali italiani Mario Staderini. Con la questione della Tirrenia, come dicevo, abbiamo un esempio dell'attuale modello di intervento pubblico in economia: la privatizzazione di una compagnia storica, che tutti noi da sempre conosciamo, specie per chi viene dalle Regioni dove questa è stata attiva. Il processo è stato avviato alla fine dell'anno scorso e prevede, come è stato ricordato nelle relazioni, la vendita separata delle società regionali Caremar, Saremar, Laziomar e Toremar e quella congiunta di Tirrenia-Siremar, il mantenimento però di situazioni di favore nella disciplina degli accosti e la concessione decennale di sussidi statali pari a 200 milioni di euro l'anno per assicurare il servizio universale. A pochi giorni dal termine previsto per il completamento della privatizzazione, la situazione è, quindi, la seguente: i bandi della società regionale sono fermi; la gara per l'acquisizione della capogruppo e di Siremar si è ridotta ad un'anomala partita a due; i lavoratori - è stato più volte ricordato anche ieri - rimangono nell'assoluta incertezza e le procedure di infrazione avviate dall'Unione

L'altro problema riguarda i 2 miliardi di euro di sussidi statali garantiti agli acquirenti per assicurare il diritto alla mobilità agli abitanti delle isole; questo problema sicuramente si porrà, come si porrà quello dei rapporti con l'Unione europea, che vieta tutta una serie di clausole che invece sono state incluse nel decreto. Siccome gli effetti di queste, nel decreto. Siccome gli effetti di queste, chiamiamole così, riforme si protraggono nel tempo e sono difficili da eliminare, occorrerà ben presto tornare ad annullare tutti i bandi, liberalizzare il settore del cabotaggio marittimo e definire con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico che si intende finanziare. finanziare. Questi possono essere i cardini intorno a cui il dibattito potrebbe essere aperto e concluso. Non so se vi sia stata concertazione tra chi ci ha presentato ieri la relazione di maggioranza e di minoranza e chi ha

allo stretto necessario, cioè allo zero. Sicuramente, per una questione come questa, che non è fondamentale per la vita del Paese, seppur molto importante per milioni di italiani, si è andati ancora una volta contro gli auspici del Colle. finestra") *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prassi parlamentare dei primissimi anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione non sembra fosse del tutto favorevole alla emendabilità dei decreti-legge. Quella stessa prassi, tra l'altro, non conosceva il malvezzo dei decreti *omnibus* il cui primo esempio, se non erro, risale al cosiddetto decretone del Governo Colombo del 1970. La stessa natura del decreto-legge come provvedimento puntuale e, quindi, essenzialmente omogeneo, così come del resto ribadito ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge n. secondo il quale «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo», dovrebbe escludere a priori la possibilità di trovarsi di fronte a provvedimenti come quelli al nostro esame. Con la sentenza n. 128 del 2008, la Corte costituzionale ha escluso la possibilità di introdurre emendamenti estranei alla *ratio* del decreto-legge. Ebbene questo potrebbe essere anche l'*incipit* di una lezione di diritto costituzionale, ma certo di una lezione un po' noiosa, tenuta in una di quelle vecchie università italiane, ormai ad un passo dal declino per lasciare il posto all'università del pensiero liberale. Allora, quanto detto sul contenuto omogeneo e sulla conseguente emendabilità di un decreto-legge non sta più in piedi. La necessità che il contenuto del decreto sia corrispondente al titolo è una pura sciocchezza, perché come criterio viene assunto lo stesso che si usa per le ricerche sulla rete, o per le banche dati, ma alla voce «ricerca semplice». Mi spiego: il requisito di ammissibilità è individuato nella presenza di una parola che ricorra identicamente sia nel titolo del decreto che nell'emendamento. Così per i fortunati che hanno già preso qualche lezione a Villa Gernetto, sede ancora in costruzione dell'università del *Premier*, trasporre il decreto sull'autotrasporto in quello sul commissariamento della Tirrenia, non è nulla di più che la prassi, trattandosi di norme che riguardano tutte il trasporto. Eppure nel titolo dell'Atto Senato n. 2262, emerge chiaramente che ciò che si cerca di garantire è il trasporto pubblico marittimo. Ed è questo aggettivo che per noi fa la differenza. Cosa hanno a che fare i vettori, i committenti, le merci, gli imballaggi, i costi minimi con la Tirrenia e la Siremar? Cosa c'entra la nomina di un amministratore unico per traghettare la Tirrenia fino al 30 settembre con l'accordo raggiunto dal Ministero delle infrastrutture con gli autotrasportatori? L'unico comun denominatore è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dunque sono obbligato a dire che forse al tavolo del Dicastero molte scelte potevano essere più ponderate. Mi riferisco alla decisione di acconsentire all'inserimento del contenuto dell'accordo con gli autotrasportatori prima nella manovra e

si trova oggi ad esaminare sì un decreto composto da un solo articolo che dispone il commissariamento della Tirrenia e della Siremar fino al 30 settembre 2010, ma non riusciamo a comprendere il senso del provvedimento in esame se non analizziamo prima il processo più generale di privatizzazione della Tirrenia.

di Tirrenia e Siremar - ossia quella presentata dalla Mediterranea Holding - ed ancora oggi Fintecna continua ostinatamente a mantenere una posizione poco chiara sull'accettazione o meno della stessa unica Viene allora da chiedersi quale sia la spiegazione logica di un tale pasticcio. Forse l'inconfessabile consapevolezza del Governo e di Fintecna che il bando di gara sia stato un fallimento? O che l'offerta di Mediterranea Holding, cordata composta dalla Regione Sicilia per il 37 per cento, che il ministro Matteoli ha frettolosamente giudicato "formalmente ricevibile", sia in realtà del tutto irricevibile? Disertata per prima proprio dai maggiori gruppi armatoriali privati, come Moby (che della contestazione alla concorrenza sleale del gruppo pubblico Tirrenia aveva fatto il proprio cavallo di battaglia), dopo la rinuncia anche del fondo americano Civen la gara è stata pressocché inesistente. Per capire meglio la vicenda, però, occorre fare un piccolo passo indietro. Alla fine del 2009, grazie ad un accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Campania, Toscana e Sardegna hanno acquisito a titolo gratuito le compagnie regionali (rispettivamente Caremar, Toremar e Saremar), passaggio considerato necessario per semplificare la procedura di gara. Unica eccezione, proprio la Sicilia, che denunciando lo stato di eccessivo indebitamento della controllata, aveva declinato l'offerta.

Resta, poi, il quesito principale: ha senso una privatizzazione che vedrebbe subentrare al controllo dello Stato quello di un ente pubblico, seppure in compartecipazione? Il senso di tutta l'operazione è forse un altro. Si tratta dei contributi pubblici che saranno ancora garantiti dallo Stato in futuro: 70 milioni per 8 anni a Tirrenia e 55 milioni per 12 anni alla Siremar. Praticamente un'altra privatizzazione all'italiana, che il Ministro giura essere al riparo dalla scure europea ma che, visti i sospetti già avanzati da Bruxelles, potrebbe dare adito a ricorsi da parte dei soggetti esclusi. A ciò occorre aggiungere che, secondo dati di inizio giugno, risultano essere ancora fermi i bandi regionali per privatizzare le società territoriali

delle linee di collegamento alle isole pontine. Eppure il cosiddetto decreto Ronchi prevedeva che la cessione del ramo d'azienda al Lazio dovesse avvenire entro il 28 febbraio 2010, data prevista per la pubblicazione del bando di gara. Per le altre due Regioni il giorno previsto per l'avvio della gara era il 31 dicembre 2009. Solo la Toscana ha pubblicato (a gennaio) il bando, ma poi si sono fatti pochi progressi. Lo stesso vice ministro Vegas, nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione lavori pubblici del Senato, ha lasciato trasparire la possibilità del non completamento della privatizzazione, che potrebbe aprire scenari fortemente critici per le società concessionarie,

convenzioni per scaduta proroga, renderebbe impossibile, a quella data, mantenere il servizio pubblico di cabotaggio. Lo stesso Vice Ministro, inoltre, ha già parlato di un possibile piano B, ossia la messa in gara delle singole linee e, quindi, la fine della società con le relative conseguenze sull'occupazione. A tutto questo, il decreto al nostro esame non dà alcuna risposta, alcuna garanzia, né sul fronte della gara, né su quello di un possibile smembramento, tanto meno sui livelli occupazionali. Siamo solo alle prese con il vostro reiterato, *ad abundantiam*, cavallo di battaglia, cioè la deroga.

in materia contenute nel codice civile, si è provveduto alla nomina di un amministratore unico delle suddette società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. C'era davvero bisogno, al fine di favorire la stabilizzazione finanziaria della Tirrenia, di far decadere l'attuale organo di amministrazione, gettando così nel caos l'azienda? Era necessario esautorare da ogni responsabilità l'amministratore unico?

riferisce dello stato di incertezza che ad oggi condiziona il buon esito della procedura di privatizzazione e che avrebbe determinato, in particolare nelle ultime settimane, notevoli difficoltà di carattere finanziario in capo a Tirrenia e a Siremar. A causa della stessa incertezza gli amministratori della società avrebbero ritenuto di non dover utilizzare anche alcune linee di credito ancora disponibili. Allora, mi chiedo se non sarebbe stato più opportuno accertare la quantità di risorse attualmente disponibili prima di chiedere nuovi finanziamenti. La nostra preoccupazione resta principalmente quella degli effetti devastanti sui livelli occupazionali. Questo mi pare al momento il punto più importante, su cui l'Italia dei Valori ha voluto presentare anche un ordine del giorno. Si vocifera il possibile fallimento dell'operazione di privatizzazione, con tutte le ricadute sociali ed economiche, ma non si tiene minimamente in considerazione il fatto che sono stati estesi già con il cosiddetto decreto-legge salva infrazioni, i meccanismi di integrazione salariale a tutto il personale in esubero della Tirrenia per un importo pari a 15 milioni per 12 mesi. Cosa accadrebbe in caso di messa a gara delle singole rotte? Cosa viene previsto per i lavoratori qualora dovesse esserci il famoso spezzatino? È più che palese il clima di superficialità e - aggiungo - di illegalità, oltre che di confusione, con cui avete operato.

e quant'altro. Poi si colpevolizza la magistratura amministrativa, quando l'errore nasce invece da queste Aule e dal fatto che non si ottempera né al dettato costituzionale né al richiamo del Presidente

esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici. Si tratta di un periodo di circa due mesi, che va da cinque giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in essere dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è posta a carico esclusivamente delle società interessate. La medesima lettera esclude negli stessi limiti la responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti citati, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Queste due disposizioni insieme, in buona sostanza, escludono ogni forma di responsabilità civile e amministrativa per gli amministratori unici nel periodo citato.

alla responsabilità dei dipendenti pubblici e al buon andamento della pubblica amministrazione. Il precedente richiamato, quello di Alitalia, addirittura estendeva l'irresponsabilità ai reati penali.

Si parla, infatti, di esclusione della responsabilità civile e amministrativa dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Considerato che sempre lo stesso comma più avanti parla di assenza di incompatibilità tra il ruolo di commissario e quello di titolare di cariche pubbliche, non si capisce il motivo di questa ulteriore specifica: e si sa che quando in una legge si scrive troppo, o si fa confusione o si vuole introdurre una norma un po' surrettizia.

la nostra Costituzione all'articolo 81 non prevede che i provvedimenti facciano riferimento ai saldi di bilancio, ormai concetto sacrale, per non parlare di entrate e di uscite.

un po' di storia. Il 23 dicembre 2009 Fintecna Spa ha avviato la procedura per la cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia e della controllata Siremar, mediante invito a manifestare interesse all'acquisto di 108.360 azioni che rappresentano l'intero capitale sociale di Tirrenia Navigazione Spa. Il bando, scaduto alle ore 12 del 19 febbraio 2010, non ha suscitato alcun interesse da parte del mercato. Vorrei ricordare che dal 1984 Franco Pecorini è l'amministratore delegato di Tirrenia Spa e che la sua gestione è stata messa in forte discussione per investimenti costosi, risultati nel tempo sbagliati, come la commessa relativa al periodo 1996-1997, che ha comportato l'acquisto di quattro costosissimi traghetti superveloci di grandi dimensioni, utilizzati per breve tempo ed ora in disuso per gli onerosi costi di gestione. Reiterati investimenti, frutto di tale inefficiente e scriteriata gestione, hanno creato di fatto una società che ad oggi è impossibile collocare sul mercato. Infatti, la flotta Tirrenia, valutata tra i 400 e i 450 milioni di euro, non vale neanche il debito, che è di circa 700 milioni. Tecnologicamente superata per il 60-70 per cento degli stessi traghetti, la flotta comprende, tra 1'altro, quattro mezzi veloci commissionati cinque anni fa a Fincantieri, ma che sono fermi da anni poiché, sebbene moderni, sono antieconomici: mezzi che appartengono ad un'era di crescita e non di crisi e che non hanno alcun valore per un mercato fortemente competitivo. Il decreto-legge in esame reca una serie di norme transitorie dirette ad assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole nel periodo di intenso traffico estivo, nelle more del completamento delle procedure di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia Spa. Infatti, come ricordato, il processo di privatizzazione di Tirrenia e della controllata Siremar, avviato da Fintecna, è in fase di avanzata realizzazione. Tuttavia, lo stato di incertezza che condiziona il buon esito della procedura nelle ultime settimane ha determinato difficoltà di carattere finanziario in capo a Tirrenia e Siremar, in presenza anche di una situazione nella quale gli amministratori della società hanno ritenuto di non utilizzare anche alcune linee di credito in essere. A tale proposito, un eventuale non completamento della privatizzazione nei tempi e nei termini previsti potrebbe aprire scenari fortemente critici per le società concessionarie, con potenziali rilevanti ricadute anche di natura economica e sociale. Così, nel caso non si riuscisse a completare la privatizzazione, il Governo avrebbe già pronto un piano alternativo che prevede la messa in gara delle singole rotte, anche se questa soluzione è la meno desiderabile poiché solo il buon esito del processo di privatizzazione potrebbe assicurare la continuità dell'attività del gruppo Tirrenia attraverso l'entrata in vigore delle nuove convenzioni. L'eventuale non completamento della privatizzazione nei termini e tempi previsti potrebbe aprire scenari fortemente critici per la società concessionaria giacché, desidero ricordarlo, l'Unione europea ha stabilito il 30 settembre come termine ultimo per l'uscita dello Stato dalla Società Tirrenia Spa. Ci auguriamo pertanto che questo possa essere il capitolo finale di una storia di marineria che, più che orgoglio, ha creato ai contribuenti pesanti oneri, visti i continui contributi che lo Stato ogni anno è stato costretto ad elargire a copertura dei clamorosi buchi di bilancio, oggi non più sostenibili.

che ha visto le parti interessate dibattere per sette lunghi mesi al fine di completare una riforma, quella della liberalizzazione regolata, introdotta sempre dai Governi Berlusconi in passato. L'accordo è stato ampio e ricalca pienamente i contenuti dei protocolli sulla legalità, trasparenza e tracciabilità che recentemente il ministro Maroni ha sottoscritto allo scopo di premiare le imprese che intendono operare nella legalità e nel rispetto delle regole. L'accordo prevede e detta disposizioni che vanno a toccare tutti i soggetti che partecipano ad un'operazione di trasporto e deliberatamente violano le norme sulla sicurezza sociale e della circolazione. Vengono, inoltre, finalmente posti limiti a coloro che da intermediari sfruttano la debolezza di tanti operatori monoveicolari ed impongono loro prezzi incompatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza. come sta facendo un intermediario che opera con una conosciuta impresa di Torino, significa costringere quell'operatore ad infrangere tutte le norme e a scaricare sui consumatori e sui cittadini incolpevoli le conseguenze messe in atto per cercare non di guadagnare, ma di perdere di meno. Con questo emendamento si creano i presupposti perché il nostro trasporto possa essere più europeo, più sicuro e più trasparente. Le norme sono chiare: nessuna limitazione è prevista per le parti che liberamente stipuleranno dei contratti di trasporto, come invece sostiene chi vuole continuare ad avere le mani libere e sfruttare la propria posizione dominante; solo la possibilità per un terzo interessato o un giudice di poter coinvolgere nelle responsabilità coloro che deliberatamente hanno concorso a violare le norme sulla sicurezza sociale e della circolazione. Tali norme non sono in contrasto con gli orientamenti europei come si apprende, in Francia per la sicurezza sono andati addirittura oltre, introducendo tariffe *antidumping*. Il Governo intende invece fissare delle regole alle quali far riferimento per poter ottenere i legittimi risarcimenti da tutti coloro i quali sarà accertata la responsabilità nella violazione delle disposizioni.

Con una battuta si potrebbe dire che allora potremmo inserire in questo disegno di legge anche un emendamento sui carri funebri, perché sempre di trasporto si tratta, o anche sugli aerei, sui treni: qualsiasi argomento riguardante i trasporti può essere inserito

il quale ho condiviso un turno pomeridiano abbastanza difficile nell'ultima seduta della Commissione bilancio in sede di esame degli emendamenti accantonati il senatore Grillo ebbe a protestare vibratamente perché, già nella manovra, si tentavano di inserire esattamente

accettabile. Nel merito, poi, di questo emendamento ci sarebbe molto da discutere, soprattutto se avessimo potuto esaminarlo con un po' più di attenzione. Per quello che si vede, la prima semplice domanda che mi pongo leggendone il testo è la seguente: dove è finito il liberismo che abbiamo (che avete) predicato per tanto tempo?

sei mesi fa, se non ricordo male, l'amministratore delegato di MSC, che è uno dei più grandi operatori marittimi del mondo, in un'interessante intervista su «Il Sole 24 Ore» consigliava caldamente al presidente Berlusconi, del quale peraltro dimostrava di essere amico e sodale, di non procedere alla privatizzazione in un momento di pesantissima crisi crisi del trasporto marittimo e dei noli come questo. Ciò, per dire che le privatizzazioni (e in questo Paese se ne sono fatte tante, alcune ben riuscite, altre francamente meno) si devono fare nel momento in cui il mercato è disposto a remunerarle, a sobbarcarsi gli oneri che spesso comporta una privatizzazione.

peccato che il maggiore azionista di tale società privata (anche se non è l'azionista di maggioranza: qui è la raffinatezza) sia un'istituzione pubblica, la Regione Sicilia. Quella stessa Regione Sicilia che aveva rifiutato qualche mese prima il regalo della Siremar.

stiamo davvero privatizzando, o stiamo assistendo a una falsa privatizzazione, cioè a una diversa forma di pubblicizzazione della Tirrenia? Questo è il primo quesito. Poi c'è un quesito ancora più angoscioso, se vogliamo: ci sono termini che vanno a scadenza in brevissimo tempo (si dice entro il 30 settembre), non non si è ancora capito che cosa ci sia nella proposta di questa Mediterranea Holding, le opinioni espresse da Fintecna non sono esaustive, si sussurra sui cosiddetti mercati con una sempre maggiore insistenza che la stessa Mediterranea Holding - che è stata buona ultima, e unica, a manifestare interesse per la Tirrenia - starebbe meditando di lasciare la partita. La domanda è molto semplice: qual è la via d'uscita, nel caso succeda questo? Qualcuno - il Governo, la Fintecna

sono state sviluppate anche considerazioni condivisibili; tuttavia, la privatizzazione della Tirrenia

in virtù della vendita o dell'acquisto di azioni sul momento, ma sono il frutto di una serie di disposizioni legislative e amministrative

Prima di arrivare a sviluppare le considerazioni sul merito del decreto, che coglie soltanto alcuni aspetti della fase finale del processo di privatizzazione, è di qualche interesse ripercorrere la storia che ha portato ai nostri giorni a queste decisioni, perché attraverso la Tirrenia si ripercorre un po' anche la storia del nostro Paese.

dopo il 1993, dopo gli accordi di Maastricht, quindi dopo l'irrigidimento necessario del bilancio dello Stato. Negli anni Ottanta nascono le società regionali. È il tempo in cui le società dello Stato diventano strumento anche di coesione sociale, e quindi strumento per la soluzione di

quegli anni. Parliamo comunque di una società che ha avuto e ha un'importanza strategica nel nostro Paese, perché sicuramente più di altre garantisce la continuità territoriale.

non abbia a diminuire la qualità e la quantità di servizio offerto da questa società, perché ne verrebbe penalizzato il sistema Paese. Alcuni requisiti sono assolutamente condivisibili, così come impostati nel processo di privatizzazione. Uno tra tutti: quello della redazione di piani industriali compatibili con il periodo di 8 e 12 anni relativo alle concessioni e alle concessioni anche di risorse pubbliche in virtù del tipo di servizio universale che viene garantito da queste società. Peraltro, sono risorse che tra Siremar e Tirrenia raggiungono, se non ricordo male, l'ordine di grandezza di 150 milioni di euro l'anno: quindi, risorse assolutamente importanti.

naturalmente di servizio. L'unica offerta che ha resistito fino alla fine - perché il 28 giugno abbiamo avuto soltanto l'offerta di Mediterranea Holding, che è stata ritenuta accettabile rispetta sostanzialmente questi requisiti. Quindi, riteniamo che sia giusto che si vada fino in fondo e si persegua l'obiettivo di arrivare finalmente alla privatizzazione della Tirrenia e della Siremar entro il 30 settembre 2010, previsto dall'impianto normativo che si è succeduto in questi ultimi anni, e in particolare dal decreto-legge 25settembre 2009, Mi sembra che il decreto-legge, presentato proprio negli stessi giorni in cui Fintecna ha ritenuto ammissibile l'offerta, vada nella direzione di garantire in quest'ultima fase il mantenimento in vita dei servizi che Tirrenia svolge e che richiedono un ultimo sforzo di natura finanziaria per arrivare alla conclusione dell'*iter*. Ci si è mossi sostanzialmente, per quello che riguarda la nomina degli amministratori, nella direzione che si era già sperimentata in altre situazioni simili (mi riferisco in particolare all'Alitalia),

In secondo luogo, è molto particolare la norma che prevede la prededuzione degli ulteriori crediti necessari da parte degli istituti finanziari, per garantire appunto la vita e la continuità territoriale dei servizi in questo periodo particolarmente delicato sia per il settore turistico, sia in generale per la mobilità nel Paese.

di un passo indietro in ordine alla liberalizzazione, perché non riapriamo i termini di negoziazione terza delle tariffe,

che non si possono stipulare contratti al di sotto di alcuni minimi rappresentati dai costi puri sostenuti dal settore. Mi sembra una norma di moralizzazione in questa fase particolarmente delicata per il settore e quindi, anche in questo caso, l'iniziativa del Governo

la Tirrenia, si è trattato soprattutto di una occasione per riaprire un sempre utile dibattito sul processo di privatizzazione in corso, illustrando alcune preoccupazioni - peraltro assolutamente condivise dalla maggioranza - per l'occupazione, per il tema della continuità territoriale, per il rispetto delle normative europee nell'ambito del processo di

e dell'attribuzione di poteri all'amministratore straordinario che sostituisce il consiglio di amministrazione, che, a parità di altre condizioni, ha certamente l'effetto di migliorare le prospettive del processo di liberalizzazione per i poteri che conferisce all'amministratore,

in buona parte fondata; io stesso ho proposto, a titolo personale - lo preciso - e quindi non come relatore e quindi impegnando la mia maggioranza, qualche emendamento in questo senso. Debbo altresì ammettere, proprio da liberale, che ci sono anche alcune ragioni contro la libertà assoluta. In primo luogo, la struttura classica ad oligopsonio del mercato a valle, cioè il mercato della logistica: gli spedizionieri e gli operatori logistici sono pochi e concentrati, hanno un grande potere contrattuale e lo sfruttano a detrimento dell'autotrasporto. In secondo luogo, la rigidità del mercato dei carburanti. E, ancora, le ragioni della sicurezza stradale, che che impongono evidentemente di non rischiare che la libera contrattazione dei prezzi porti a ridurre le condizioni della sicurezza. Va poi detto, come ricordato dal senatore Cicolani, che non si tratta proprio di un ritorno a tariffe obbligatorie, ma semplicemente di stabilire un minimo che consenta di non mettere a rischio le condizioni della sicurezza della circolazione. Un mio emendamento concentra il tema della tariffa minima proprio sul vettore che materialmente effettua il trasporto, saltando gli intermediari che spesso ci sono in questa industria e che non hanno in questo senso particolare motivo di godere di agevolazioni di questo tipo. Questo è quanto mi pareva utile ribadire nel merito, ringraziando tutti gli intervenuti nella discussione generale,

Signor Presidente, signori senatori, sulla Tirrenia sono stati esaurienti sia l'intervento del senatore Cicolani che quello

Stiffoni, vorrei dare una risposta ad un senatore a cui mi lega un'amicizia antica, il senatore Sircana,

Il tema dell'autotrasporto è fondamentale per la nostra economia. A causa delle politiche di trasporto e delle infrastrutture degli ultimi 30 anni, cento dei trasporti del nostro Paese si svolge su gomma. Questo definisce il ruolo dell'autotrasporto e del trasporto su gomma Questo definisce il ruolo dell'autotrasporto e del trasporto su gomma come molto più che essenziale. Vede, senatore Sircana, c'è un punto

far cessare un blocco dei TIR che durò giorni e giorni, adottò dei provvedimenti molto più severi di quelli di cui discutiamo in questo emendamento. Il Governo Prodi,

tra i quali - altro che controriforma dell'autotrasporto! - le tariffe *antidumping*, che sono il contrario della liberalizzazione adottata in questo Paese nel 2005. Il punto è che in questa legislatura Il punto è che in questa legislatura l'autotrasporto è stato toccato da due crisi pesantissime: l'aumento del costo del gasolio e la crisi economica più grave del dopoguerra.

Abbiamo detto che l'autotrasporto italiano ha un eccesso di offerta che lo indebolisce rispetto alla committenza.

dai vari Governi con l'autotrasporto: il risultato di tali politiche e di tali intese (tra cui quella del Governo Prodi del 2007) è che, vent'anni dopo, ci troviamo ad dei trasporti su gomma, con un eccesso di offerta e con una domanda in grado di determinare le condizioni. Nell'ultimo accordo, del 1° dicembre 2009, il Governo ha cercato una strada nuova: ha, cioè, detto di non voler più calare l'accordo tra Governo e autotrasporto nel mercato, ma di voler organizzare un tavolo di confronto a tre, a cui partecipassero Governo, autotrasporto e committenza.

Con l'accordo del 17 giugno - senatore Sircana - per la prima volta noi non soltanto evitiamo il blocco dei TIR al Paese,

luogo, nei prossimi sei mesi noi prepareremo il nuovo piano della logistica, all'interno del quale componente fondamentale sarà la politica industriale del settore, che punta a ridurre la frammentazione e ad agevolare e incentivare le aggregazioni, per consegnarci un settore più forte e competitivo, non soltanto per l'industria italiana, ma anche per il mercato europeo. abbiamo costituito un gruppo fatto di esperti giuristi dei trasporti, con i quali poniamo mano a un lavoro

all'esame e al dibattito del Parlamento e delle Commissioni parlamentari. Per questi motivi, ritenendo di aver fatto l'interesse del Paese e non del Governo, avendo difeso in questi due anni un settore strategico per la nostra economia come quello dell'autotrasporto, chiedo il voto favorevole su questo provvedimento.

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.100 e i relativi subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

di fatto determina alcuni elementi di particolare apprensione dal punto di vista occupazionale per l'indicazione degli elementi a carattere numerico indicati (vale a dire le 196 unità per la Tirrenia e le 15 unità per la Siremar),

pochi emendamenti presentati, per rendere coerente l'impianto normativo del provvedimento al suo titolo originario.

suddette. L'emendamento 1.5 è volto a ricostituire le responsabilità civile, amministrativa e contabile dell'amministratore unico, peraltro già nominato dal momento che il decreto-legge, oggi in conversione, è di fatto già effettivo.

è la reale finalità per cui si giustifica tale provvedimento straordinario, e non altro. Altrimenti avremmo davvero creato un *killer* con la licenza di uccidere senza alcuna responsabilità, la quale ovviamente ricadrà su chi poi rileverà le due società di gestione.

Mi dispiace che non sia presente in Aula perché, dovendo parlare di una sua decisione, avrei preferito farlo in sua presenza. L'emendamento che è stato dichiarato ammissibile non ha nulla a che vedere con il provvedimento che stiamo esaminando. una materia totalmente estranea alla questione.

la navigazione nelle acque nazionali del nostro Paese, non regolamenta il servizio, non regolamenta la flotta, non regolamenta le frequenze, non regolamenta nulla. Riguarda soltanto l'amministratore unico.

Ha un valore che va anche al di là dello stesso merito del problema che si sta esaminando? Penso di sì. Penso che ieri, di fronte alla richiesta molto chiara e reiterata dal senatore Legnini, il presidente Schifani abbia adottato una decisione di carattere politico, di carattere esclusivamente politico. Davanti alla richiesta del Governo, che chiedeva di inserire in questo provvedimento un emendamento che aveva già cercato

davanti a questi tentativi non riusciti, il Governo prende un vagone in transito, finge che vi sia una connessione e inserisce e inserisce l'emendamento in un provvedimento estraneo. Con la sua decisione il presidente del Senato ha sostanzialmente dato

può servire per far passare una norma nel modo irrituale in cui accade oggi con questo emendamento, il Governo dispone ed il Senato esegue.

che riguarda noi, che riguarda il tema che abbiamo più volte sollevato della funzionalità e dei modi della funzionalità del lavoro del Senato. Perché questa decisione pesa negativamente sui nostri lavori? Innanzitutto, è una decisione che, in qualche modo, influisce sui rapporti dell'opposizione con la maggioranza e, mi dispiace doverlo dire, anche con la Presidenza dell'Assemblea.

Il nostro Regolamento - ed io concordo - attribuisce al Presidente del Senato dei poteri discrezionali molto consistenti. Ma questi poteri discrezionali sono attribuiti al Presidente per garantire i lavori dell'Assemblea e debbono essere a mio parere (e ripeto posizioni già espresse) esercitati con una particolarissima attenzione quando si tratta di decidere su questioni riguardanti l'interesse politico del Governo e le posizioni rigorose dell'opposizione nella interpretazione del nostro Regolamento. Quando ieri ha preso la parola il senatore Legnini illustrando le ragioni dell'inammissibilità, non ha replicato al senatore Legnini il relatore, non ha replicato il Governo, non è intervenuta la maggioranza: è intervenuto il Presidente, che ha chiuso lì la questione. Questo, a mio parere, è un modo di il lavoro del Parlamento, l'insieme delle nostre regole e delle nostre prassi, la gestione gelosa dei precedenti che fa l'amministrazione del Senato (che noi non conosciamo e di cui non abbiamo la possibilità di disporre). È questione che non viene sollevata dall'opposizione: che finora non viene sollevata dall'opposizione. però, non viene sollevata nel presupposto che la Presidenza utilizzi questo suo deposito di sapere in un modo equidistante: non voglio dire che protegga l'opposizione in quanto minoranza e, quindi, e, quindi, con un maggior bisogno di protezione. Guardate, qui è in gioco la sostanza della democrazia parlamentare. Questo è il vero problema. Ed è in gioco anche la qualità della legislazione, alla quale più volte il Presidente della Repubblica ci ha richiamato. Io considero la decisione di ieri del Presidente del Senato un decisione politica e non tecnica - l'ho già detto - e considero che a questa decisione siano stati estranei i pareri tecnici dell'amministrazione del Senato. Escludo che l'amministrazione del Senato abbia potuto consigliare il Presidente in modo decisivo, dando un'interpretazione tecnica dei Regolamenti. Questa è stata una decisione politica. danni di queste decisioni sono, a mio parere, molto consistenti. Il nostro lavoro si regge su un equilibrio molto delicato, che è fatto di misura nelle decisioni. Io non entro nel merito del provvedimento, signor Presidente, ma entro soltanto nella questione del rispetto delle regole e della necessità

la condivisione e il sostegno al ragionamento articolato, puntuale e preciso del collega Zanda. Ancora una volta, l'attività legislativa del Senato viene turbata, oserei dire violentata, dall'inserimento in un provvedimento di norme che con lo stesso provvedimento non hanno niente a che vedere. E poiché i richiami del Capo dello Stato non possono essere utilizzati a senso unico, a senso unico, ma sempre considerando quello che egli ci dice dall'alto del magistero costituzionale, vorrei ricordare che

È chiaro che vi è stata una forzatura, a nostro avviso un errore nel procedimento legislativo; ecco perché invitiamo la Presidenza non assumersi più responsabilità di questo tipo, che sono gravi e certamente, queste sì, turbano il corretto e leale andamento dei lavori parlamentari.

la parte svolta in Commissione bilancio quando, avendo letto un emendamento che a parer mio non aveva nessuna relazione con una manovra finalizzata a contenere i costi e a ridurre le spese, ho avuto modo, assumendomene la responsabilità nella mia qualità di Presidente della Commissione di merito, di criticare questa procedura, così come è avvenuto - lo sanno i colleghi dell'8a Commissione - tutte

della possibilità di gestire e governare questo parere. Tutto ciò premesso, però, ritengo che sia il collega Zanda sia il collega Belisario abbiano un po' enfatizzato questo passaggio. Lo dico perché, a mio modo di vedere, dicendo le cose che sono state dette si ignorano alcune questioni. Certamente anche a noi membri della Commissione sarebbe piaciuto che questo emendamento venisse presentato in Commissione, magari dopo l'approvazione di un decreto *ad hoc* da parte del Governo, siamo al 21 luglio e un decreto emanato in questi giorni avrebbe fatalmente corso il rischio di non essere convertito entro i fatidici 60 giorni,

obiettivo: quello di evitare il blocco dei TIR in questi due anni, che saranno, secondo la nostra opinione, due anni difficili, di possibile, sperata ripresa economica, in un Paese che trasporta il 90 per cento della merce, e quindi della produzione,

che rappresentano gli operatori dell'autotrasporto: è un altro risultato che noi ascriviamo in positivo ai meriti del Governo. Certamente, se si chiede a noi, che abbiamo in questi anni seguito il processo evolutivo iniziato nel 2005 con il decreto che ha liberalizzato il settore, se queste norme che sono un poco più garantiste nei confronti degli operatori del settore rappresentino un passo avanti o un passo indietro nella logica di un mercato sempre più

essere stata coscientemente voluta e sottoscritta dal Governo data la crisi del contesto generale. Mi consentirà il senatore Zanda di riprendere un'osservazione, acuta, del senatore Sircana, quando, riferendosi a quanto detto dall'amministratore delegato di MSC, si chiede: ma sono ora i tempi maturi, giusti, appropriati per insistere su questi processi di privatizzazione, oppure dobbiamo tenere conto dei rischi che si nascondono in questo contesto, attorno a questa decisione? Non c'è dubbio: dobbiamo essere realisti, tenere i piedi per terra. L'Europa ci dice che le liberalizzazioni vanno fatte: il procedimento

in assoluta coerenza e sintonia. Siamo arrivati, dopo 16 offerte di possibili acquirenti della Tirrenia, ad un solo acquirente, il quale ha presentato un piano industriale che peraltro

in una sorta di dialogo competitivo - sia possibile migliorarlo ed integrarlo, soprattutto nella prospettiva di dare maggiori garanzie ai livelli occupazionali esistenti, al patrimonio vero che Tirrenia ha costruito in questi 30‑40 anni di operatività.

esprimere un giudizio sulla prepotenza - se esiste - della maggioranza, che umilierebbe l'Aula imponendo un emendamento che nessuno conosceva. Questo emendamento, sia detto per inciso (ma non lo dico io,

noi voteremo contro questa ipotesi emendativa, per le motivazioni che poco fa ho ricordato.

il senatore Latorre ieri ha partecipato, come me, alla Conferenza dei Capigruppo, dove l'argomento che stiamo affrontando è stato menzionato.

della questione si è parlato in Conferenza dei Capigruppo, si è comunque convenuto. Io stesso ho avuto ulteriori contatti con esponenti della minoranza, che avevano piena consapevolezza di questo modo di procedere, che noi riteniamo corretto e rispettoso delle regole, nella

sia un provvedimento congruo. Immagino, senatore Zanda, che se non ci fossero stati provvedimenti sull'autotrasporto, stando all'opposizione - condizione vantaggiosa per certi versi - lei si sarebbe alzato e con la stessa enfasi avrebbe detto: questa maggioranza e questo Governo non fanno nulla per affrontare il blocco dell'autotrasporto, che penalizza gli italiani in piena estate, con le code delle vacanze sulla Salerno-Reggio Calabria. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Potrei fare io al suo posto - ma non posso sostituirla, non sono alla sua altezza - l'intervento che lei avrebbe fatto per protestare per il blocco dell'autotrasporto: «L'autotrasporto non si blocca!» La Presidenza ha operato correttamente.

al sottosegretario Giachino: «L'Autorità è ampiamente consapevole della specificità del settore dell'autotrasporto e, in particolare, del fatto che il confronto competitivo non debba non debba avvenire a scapito del pieno rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. L'Autorità ritiene tuttavia che (...) l'individuazione di "costi minimi di esercizio,"» - quindi, non si citano le tariffe minime non costituisca uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio ma piuttosto per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità. L'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori che la legge attribuisce alle amministrazioni pubbliche competenti, eventualmente rafforzato, consente di rispettare gli standard qualitativi minimi e l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di previdenza, senza la necessità

venuta meno, chiedendo, signor Sottosegretario, la possibilità di condividere il percorso che ha seguito il Governo per due ordini di motivi. In primo luogo, volevamo conferire in qualche modo una cornice e anche una articolazione di strumenti normativi che non cogliessero soltanto la specificità dei costi minimi di esercizio ma che sostanzialmente rafforzassero quel potere di controllo che è richiesto proprio dai soggetti dell'autotrasporto per applicare le norme che già esistono. il paragone con il Cile, sia da un punto di vista storico e temporale, sia perché siamo inseriti in un contesto comunitario che ha ben altre regole, sia perché oggettivamente un po' tutti - ma, consentitemi, in particolare voi - abbiamo contribuito ad una debolezza, ad una fragilità e di conseguenza ad una forza che l'autotrasporto esercita sul sistema della logistica e del trasporto merci che davvero imporrebbe ben altri strumenti, ben altre attenzioni, ben altre strategie. quindi un appello, proprio per non lasciare niente di intentato, per far capire che non c'è nessuna volontà o pregiudizio rispetto alla norma ma la necessità di condividerne il percorso, di inserirlo in una cornice normativa più organica e adeguata, e soprattutto anche per recuperare una titolarità della Commissione

che davvero - spero e mi auguro - voglia vedere rispettati, non dico pedissequamente e rigorosamente, ma almeno in termini accettabili i canoni ordinari dell' *iter* legislativo. relatore, faccia uno sforzo di coraggio, ne ha già fatti molti; abbiamo apprezzato la sua audacia ed il suo coraggio e ci dispiace che siano stati ritirati emendamenti di grande qualità che avremmo sicuramente apprezzato e votato. È un'ultima invocazione, fate voi.

dopo le parole «trasporto marittimo», aggiungere, in fine, le seguenti: «ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti»

il mio intervento sarà breve, perché l'Italia dei Valori non può essere che contraria a questo provvedimento, per il merito e, concedetemi, anche per il metodo. Ci avete abituati ormai a questo malcostume dell'attività legislativa, ad operazioni di trasposizione legislativa che stanno diventando nel corso di questa legislatura un *modus operandi* ricorrente: ma il ripetersi di questa prassi è sempre meno accettabile sotto il profilo costituzionale, normativo e regolamentare. Le Assemblee parlamentari vengono - di fatto - espropriate della funzione legislativa, e poi ci si mette anche la decisione di ieri del presidente Schifani, giustamente rilevata dal presidente Belisario. Colgo l'occasione per chiedere alla Presidenza che siano resi disponibili i precedenti relativi ai casi nei quali un decreto-legge è stato trasfuso in un altro decreto-legge, con la motivazione che entrambi erano stati adottati dal medesimo Ministero; in generale, sia messo a disposizione di tutti i Gruppi il massimario dei precedenti, come già richiesto dal senatore Belisario in occasione dell'esame del decreto-legge sugli enti lirici; sia infine investita la Giunta per il Regolamento

Dopo i fuochi d'artificio della proposta di modifica all'articolo 41 della Costituzione al fine di introdurre maggiore libertà di impresa, dopo la «paghetta» discrezionale alle comunità giovanili, siamo arrivati forse alla notizia più eclatante, signora Presidente e colleghi: quella che riguarda gli accordi sui costi minimi di esercizio e i tempi coattivi di pagamento dei trasportatori. Comparsa prima in alcuni emendamenti della manovra, poi in un decreto-legge adottato nella seduta del 16 luglio 2010 del Consiglio dei ministri e ora trasfusa nel decreto-legge Tirrenia, questa riforma della disciplina dell'autotrasporto ci è stata imposta dall'alto, nella fretta di approvarla prima della chiusura dei lavori del Parlamento e, soprattutto, prima di un nuovo sciopero degli autotrasportatori. Non è così, cari colleghi, che si risolvono i problemi del nostro Paese. Nel merito del decreto-legge vertente sulla Tirrenia e sulla Siremar, ho già detto tutto e non posso che ribadire che non c'è nulla di più confuso di questo processo di privatizzazione e di questo provvedimento. Come sempre, a pagare saranno i lavoratori.

Tirrenia è uno dei maggiori operatori italiani nel settore del cabotaggio e svolge un ruolo importante nell'economia del Paese con l'esercizio di un'attività di servizio pubblico di collegamento con le isole maggiori e minori. Se si considerano circa 6,7 milioni di residenti nelle isole maggiori, l'Italia risulta il Paese europeo con il più alto numero di abitanti in aree del territorio nazionale separate dal mare: così, la flotta cabotiera costituisce parte essenziale del sistema nazionale dei trasporti. Fino ad alcuni mesi fa, facevano parte del gruppo Tirrenia anche le società regionali dell'azienda (oggi gestite dalle Regioni competenti, salvo la siciliana Siremar): Caremar, che gestisce i collegamenti con Capri, Ischia, Procida, Ponza e Ventotene; Saremar, che si occupa dei collegamenti con Corsica, La Maddalena e San Pietro; Toremar, che gestisce i collegamenti con Elba, Giglio e Capraia. L'attività di servizio è svolta da tutte queste società in conformità a sei identiche convenzioni stipulate con lo Stato di durata ventennale, con decorrenza dal 10 gennaio 1989. A fronte dei servizi resi in regime di servizio pubblico, lo Stato corrisponde annualmente alle società del gruppo una sovvenzione di equilibrio affidati, senza gara, secondo gli obblighi di servizio pubblico, con l'obiettivo di tutela della continuità territoriale. Tirrenia però deve essere privatizzata. Lo dice il Governo, lo impongono le direttive comunitarie e il mercato: non ha senso mantenere in vita, grazie alle sovvenzioni di equilibrio (cioè gli aiuti di Stato), una società che opera in un settore che di fatto è già liberalizzato. Infatti, dopo gli accordi di programma per la regolamentazione dei servizio pubblico di cabotaggio marittimo, i consiglieri di Fintecna hanno deliberato la procedura, mediante l'invito a manifestare interesse entro il 19 febbraio, volta alla privatizzazione di Tirrenia inclusa la Siremar. Al 19 febbraio, Fintecna ha comunicato che le manifestazioni di interesse all'acquisto di Tirrenia-Siremar pervenute sono state sedici. La procedura, però, ha previsto che il consulente finanziario e il consulente legale verifichino la rispondenza ai requisiti. Così, dopo questa verifica, il numero si è dimezzato ed è sempre più reale il rischio che la privatizzazione di Tirrenia si trasformi in un *flop*: c'è chi dice che alla fine si ritireranno tutti i pretendenti e che per l'acquisto della compagnia pubblica sarà necessario bandire una nuova gara. Infatti, la presenza della Siremar, con un indebitamento finanziario di 91,8 milioni al 2008 ed una flotta composta da 19 unità, grava sulla appetibilità dell'operazione, oltre al concetto che normalmente non si cede un'azienda durante un periodo di crisi economica. La stessa Commissione europea, inoltre, ha chiaramente affermato che il sistema di convenzioni pubbliche ai vettori marittimi può giustificarsi soltanto in riferimento a quelle linee, come quella relativa ai collegamenti con le isole minori, in cui il servizio non può essere svolto adeguatamente da imprese private. Malgrado ciò, il Governo non ha voluto prevedere il blocco del processo di privatizzazione della Siremar, attraverso lo scorporo dalla privatizzazione dalla Tirrenia, con il conseguente avvio, presso l'Unione europea, del processo di deroga alla privatizzazione e quindi a dotare la nuova Siremar di un adeguato sostegno finanziario a carico dello Stato e delle Regioni, in base al principio che le ragioni di economia relativa alla spesa pubblica non possono valere nel caso di servizi così essenziali senza che nessuno intervenga in sostituzione. Signora Presidente, a nostro parere è un errore vendere ora e con questo assetto la Tirrenia. Pertanto, il voto del nostro Gruppo Signora Presidente, onorevoli colleghi, gentile sottosegretario, non è certo oggi che scopriamo che il gruppo Tirrenia è una delle principali realtà nel settore del cabotaggio marittimo nazionale. Ricordiamo che opera i collegamenti tra il continente e le due isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, e attraverso la controllata Siremar garantisce i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori della Regione. L'attività del gruppo Tirrenia ha consentito per decenni di assicurare la continuità territoriale nazionale, garantendo il servizio di pubblica utilità tramite una convenzione con lo Stato, che in questi anni ha garantito alla stessa Tirrenia trasferimenti erogati a titolo di corrispettivo per il servizio pubblico svolto, trasferimenti che nel 2009 sono ammontati a circa 210 milioni di euro. Completo questa mia breve premessa ricordando che Tirrenia di Navigazione Spa è una società controllata da Fintecna Spa (a sua volta interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze); a sua volta Tirrenia detiene l'intero capitale sociale di Siremar. Ma arriviamo ad oggi, partendo precisamente dal 23 dicembre 2009, quando Fintecna Spa avvia la procedura per la cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia. Si arriva quindi al decreto-legge all'attenzione oggi del Senato, che reca una serie di norme transitorie, dirette ad assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole nel periodo di intenso traffico estivo,

La principale finalità del decreto-legge consiste, pertanto, nel garantire la situazione finanziaria della Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso. Entrando nel merito del provvedimento, alla lettera *a)* dell'articolo 1 è prevista la nomina di un amministratore unico delle società Tirrenia di Navigazione Spa e Siremar Spa, a cui sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

sottolineare un aspetto importante: la società è stata capitanata dal lontano 1984 dall'amministratore delegato Franco Pecorini;

criticata e i risultati sbagliati hanno determinato le condizioni per cui si è arrivati ad una società di difficilissima collocazione sul mercato.

A seguito di questo decreto-legge, dalla scorsa settimana c'è un uomo di fiducia dell'azionista Fintecna alla guida di Tirrenia: è Giancarlo D'Andrea, già nell'IRI, già presidente di Alitalia Servizi, quando la compagnia di Stato andava verso la privatizzazione, e già direttore generale della stessa Fintecna. Dopo aver riassunto il processo di privatizzazione, passiamo ora ai 16 soggetti i quali, nel febbraio scorso, avevano fatto pervenire a Fintecna Spa una manifestazione di interesse all'acquisizione della società. Alla fine di giugno, c'era invece un'unica offerta di acquisto da parte di Mediterranea Holding di Navigazione Spa, Spa, società partecipata per il 37 per cento dalla Regione Sicilia, e che vede la presenza di imprese operanti nel settore armatoriale e del trasporto marittimo. La situazione può apparire strana e magari lo è, ma può considerarsi normale

A tale proposito, un eventuale non completamento della privatizzazione nei tempi e nei termini previsti potrebbe aprire scenari fortemente critici per le società concessionarie,

L'operazione di privatizzazione di Tirrenia e Siremar da parte di Fintecna registra fattori di particolare complessità in ragione, fra l'altro, della dimensione della società oggetto di vendita,

Come Lega Nord ci auguriamo che l'operazione di privatizzazione della Tirrenia si possa concludere rapidamente (penso che questo sia l'auspicio di tutti), senza ulteriori oneri per il contribuente derivanti dai continui contributi che lo Stato ogni anno è stato costretto ad elargire a copertura dei clamorosi

come sostenuto da chi mi ha preceduto, si tratta di un intervento per la sicurezza dei cittadini che garantisce trasparenza, tracciabilità e rispetto delle regole. Si possono così sintetizzare

che recentemente (come ricordato dal collega Stiffoni) il ministro Maroni ha sottoscritto allo scopo di premiare le imprese che intendono operare nella legalità e nel rispetto delle regole. regole. In questi emendamenti si creano i presupposti perché il nostro trasporto possa essere più europeo, più sicuro e più trasparente.

6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo»), pur comprendendo le ragioni delineate nell'oggetto del provvedimento non si è potuto esimere dal valutare la non effettiva rispondenza del contenuto delle norme alle finalità espresse in titolo. Come pure indisgiungibile è un giudizio di merito su siffatto provvedimento da una valutazione più complessiva sull'intero processo di privatizzazione intrapreso con riguardo alla compagnia di navigazione Tirrenia e alle compagnie di navigazione regionali ad essa collegate. A complicare ulteriormente la situazione è poi intervenuto l'emendamento del Governo, già oggetto di decreto-legge, frutto di recepimento di accordo tra le parti ed inerente ad aspetti salienti della regolamentazione dell'autotrasporto nel nostro Paese,

Rileviamo che a niente sono valsi gli emendamenti che abbiamo presentato, pochi ed essenziali, esclusivamente finalizzati a ricondurre il provvedimento in questione ad una più rigorosa osservanza della sua dichiarata finalità, quella cioè di garantire in questa fase delicata di chiusura del processo di privatizzazione il mantenimento di linee di credito finalizzate esclusivamente all'esercizio dei collegamenti di trasporto da e verso le isole del nostro Paese. modo, dispiace che a niente siano valsi anche i reiterati tentativi, svolti prima in Commissione e poi in Aula (ieri, ma anche oggi), di chiedere una sede più appropriata per recepire i contenuti di quell'accordo sull'autotrasporto siglato tra Governo e alcune categorie, inserendolo però in una cornice normativa più organica ed adeguata, anche prefigurando la disponibilità da parte nostra ad accogliere la richiesta di procedure abbreviate di approvazione. tutto ciò ci fa dire che, almeno nella sostanza, avete perso un'occasione di dialogo e di condivisione che vi era stata offerta e che avete invece sdegnosamente rifiutato tirando dritto per la vostra strada, forti nei numeri, ma davvero deboli nelle argomentazioni. Nella sostanza prendiamo atto di un'azione di governo, in questo settore dei trasporti, ormai logora, che si caratterizza per un procedere a tentoni, facendo volutamente una gran confusione tra liberalizzazioni ed apertura dei mercati, con provvedimenti discutibili di privatizzazione i cui effetti non tarderanno purtroppo a rivelarsi per ciò che sono. Il provvedimento di privatizzazione di Tirrenia, come ricordava ieri nella relazione di minoranza il collega Vimercati, nasce infatti sotto la voluta mistificazione di direttive e richiami dell'Unione europea, rivolte in realtà a ben altri obiettivi. L'Unione europea non ci ha mai chiesto di privatizzare la compagnia di navigazione Tirrenia, semplicemente perché non ce lo può chiedere. Ha chiesto un'altra cosa che rientra nelle sue prerogative e nei suoi obiettivi strategici condivisi da tutti i Paesi ad essa aderenti, quella cioè di aprire un mercato che risulta caratterizzato per certi versi da un monopolista pubblico di Stato e per altri dallo stesso soggetto pubblico in posizione dominante per determinati servizi rispetto agli altri soggetti privati, configurando per il nostro Paese una indebita azione di aiuti di Stato nella copertura dei servizi erogati. Per risolvere questa non accettabile condizione, l'Unione europea ha chiesto che venissero indicati espressamente quei servizi universali di continuità territoriale e che a garanzia dei quali fosse quantificato il necessario corrispettivo. Non certo l'Unione europea desiderava e chiedeva quello che ancora una volta, dopo la nefasta operazione Alitalia, state facendo, ossia sostituire un monopolista pubblico con uno privato o parapubblico, come nei fatti risulta essere la compagnia di navigazione Mediterranea Holding. Singolare - giusto per usare un educato eufemismo - è risultato poi il processo di vendita della compagnia di navigazione e dei servizi relativi. Infatti, dopo la manifestazione di interesse da parte di 16 soggetti imprenditoriali, a seguito della conseguente procedura di *due diligence*, un solo soggetto ha presentato un'offerta irrevocabile e giudicata congrua da Fintecna. I motivi di tali rinunce sembrano rinvenibili - come dichiarato dall'armatore greco, autorevole esponente della cordata rimasta in gara, e peraltro mai smentito - nella - nella pesante situazione debitoria emersa dalla *data room*, stimata in oltre 500 milioni di euro. Appare pertanto insolito che la Regione Sicilia, principale azionista con il 37 per cento delle quote della Mediterranea Holding, sia rimasta interessata al rilevamento della compagnia di navigazione Tirrenia e di quella regionale Siremar, con lo stato di indebitamento che ho testé rappresentato, dopo aver manifestato precedentemente la sua indisponibilità a rilevare gratuitamente la sola compagnia di navigazione regionale Siremar, per garantirne il processo di privatizzazione come parallelamente stanno facendo le altre Regioni interessate. E davvero sinistre sono suonate le affermazioni del vice ministro Vegas nelle sue apprezzabili audizioni di Camera e Senato presso le Commissioni di merito, in cui ha serenamente dichiarato che se la procedura di vendita fallisce il Governo intende procedere con il piano B, ossia con lo spezzatino, come si usa dire in gergo. Vale a dire, quindi, con la messa sul mercato delle singole rotte e dei singoli servizi, con buona pace dei livelli occupazionali

ma soprattutto con buona pace degli utenti più deboli, i residenti delle piccole isole, ai quali dovrete spiegare la loro condizione di sfigati cittadini di serie B, in uno Stato da tempo non più uguale per tutti e che oggi, con questo Governo, non si pone più neppure il problema della sua continuità territoriale e della relativa salvaguardia dei diritti sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Come pure dispiace non vedere una strategia per il Paese in un settore tanto delicato e vitale come quello dell'autotrasporto, in cui ben altro avrebbe dovuto essere il respiro riformatore di regolazione del mercato e ben altra la prospettiva di sviluppo da perseguire per quel nevralgico settore della logistica. Invece, tra Governo e categorie,

sistematicamente rilancia sul precedente senza neppure verificarne lo stato di attuazione, né valutare le effettive implicazioni di quello che lo sostituisce. Siete ridotti a giocatori di poker che, passando di rilancio in rilancio, sperano che nessuno venga mai a vedere le vostre carte. Quello che vi proponevamo era nient'altro che la condivisione di una strategia per il Paese, che fosse in grado di correggere la deregolamentazione conosciuta in questi anni dal settore dell'autotrasporto, che tante distorsioni ha generato e che costituisce una grave insidia per il sistema Paese, per un maggiore riequilibrio modale e per una migliore sostenibilità, sia ambientale che sociale, dal punto di vista della sicurezza e del congestionamento urbano e stradale. Ciò che vi proponevamo non era la semplice individuazione dei costi minimi o della tariffa minima, che nega in principio il concetto di liberalizzazione e di apertura regolata dei mercati, quanto un ventaglio di riforme in grado di dare, in una prospettiva certa, un equilibrio strutturale al settore. Ci si aspettava provvedimenti che, grazie a leve ed incentivi fiscali, fossero in grado nel breve e medio periodo di produrre quell'indispensabile processo di concentrazione di soggetti imprenditoriali la cui attuale polverizzazione è ben lungi dal costituire affermazione di libera imprenditoria ma piuttosto di deregolamentazione selvaggia, sfruttamento inaccettabile della forza lavoro e ricatto occupazionale. Quello che vi proponevamo era l'intensificazione dei controlli, non a caso chiesti *in primis* dagli stessi operatori del settore, per frenare forme di concorrenza scorretta, inaccettabile e pericolosa per l'incolumità delle persone, cosa che purtroppo non avete fatto. Forse avete avuto ragione voi a declinare l'invito che vi è stato reiteratamente offerto. Per accoglierlo, occorreva avere, almeno per il settore del trasporto delle merci, una visione chiara dello sviluppo che si vuol perseguire per il Paese. Cosa che purtroppo non avete, né è ragionevole pretendere, perché non avete neppure in animo di perseguire, come ormai attesta il vostro atteggiamento schizofrenico nell'affrontare una crisi economica di queste proporzioni. Un giorno drammatizzate la situazione per chiedere iniqui sacrifici. Il giorno dopo la crisi è già risolta e il peggio è subito alle spalle, alle vostre spalle. La credibilità di un Governo e della maggioranza che lo sostiene non è merce che si trova in commercio di questi tempi. Ed in fondo è per questi semplici motivi che non possiamo che prendere le distanze da provvedimenti mal confezionati, che risultano inaccettabili prima ancora che nel merito, per un metodo ed un modo di fare che non può appartenerci. Conseguentemente il nostro sarà un voto contrario.

l'Unione europea da più di 10 anni insiste sulla necessità e, quindi, sull'obbligo di liberalizzare l'intero settore del cabotaggio marittimo.

la realtà del mercato e dei fatti che ci obbliga a procedere lungo questa strada, sperando di trovare degli interlocutori validi, che sappiano, nel tempo, non umiliare il cospicuo patrimonio di persone

doveva concludersi il processo di privatizzazione era appunto il 30 settembre 2009 e con ciò si è dato spazio alla vendita e alla privatizzazione di alcune società controllate da Tirrenia, come la Caremar, con un'operazione che ha interessato sia la Campania sia il Lazio. Siamo poi arrivati al bando poi arrivati al bando della Fintecna, bando che ha inizialmente suscitato l'interesse di ben 16 gruppi, tra fondi comuni e società italiane ed estere. Purtroppo,

come forse ogni tanto immagina il Presidente di quella magnifica Regione, che la Sicilia possa diventare la più grande piastra logistica del Mediterraneo per i traffici di passeggeri. Evidentemente, però, io non ho interlocuzione con il presidente Lombardo e non posso fare

che stabilisce che i finanziamenti che le banche daranno per continuare la gestione corrente, in caso di - possibile, non auspicabile - fallimento, andranno in pre-deduzione: quindi le banche, sentendosi garantite, certamente offriranno ancora fidi, l'ossigeno necessario a far sì che Tirrenia vada avanti. La parte più importante non è aver nominato un commissario, che anche a me sembra

Sul punto, vorrei dire la mia opinione, che è la seguente. Rispetto l'*Antitrust*, che è una istituzione che nel tempo ha acquisito credibilità,

delle leggi), nel decidere non possiamo ignorare la realtà nella quale in questo momento vivono il Paese, il settore del cabotaggio, la realtà della Tirrenia, con il rilevante carico di dipendenti, nei confronti dei quali credo abbiamo fatto bene ad approvare gli ordini del giorno che ne auspicano la tutela, di tutti, compresi quelli che il vice ministro Vegas, nella sua pregevolissima relazione, dice che sono a rischio. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e tenere presente quanto diceva il Sottosegretario quando parlava di possibile blocco, di possibile crisi, di una condizione estremamente difficile in cui si sarebbe venuto a trovare il nostro Paese nel caso non avessimo dato una risposta normativa ad un accordo sottoscritto dalle parti. È per questi motivi, signora Presidente, che il Gruppo del PdL conferma il voto favorevole alla conversione del decreto-legge.

in particolare le Commissioni 5a e 10a, impegnate nell'esame del decreto-legge recante misure urgenti in materia di energia, all'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna, cosicché la discussione del provvedimento possa iniziare in Aula nei tempi stabiliti.

Ovviamente, la situazione è molto complicata per queste famiglie, visto che la cassa integrazione è prevista per tutto l'anno in corso. Pertanto, l'interrogazione è di per sé urgente, però volevamo sottolineare la questione all'Aula proprio per la necessità di intervenire in tempi molto rapidi.

Signora Presidente, anch'io desidero annunciare un'interrogazione su una questione che richiede un intervento molto urgente. In un Comune della Provincia di Ferrara, si è riaperto un pozzo da cui continuano ad uscire acqua metanosa e metano allo stato gassoso. Il sindaco del Comune di Berra, insieme al prefetto di Ferrara, ha chiesto un intervento all'unità locale regionale del Ministero dello sviluppo economico, che è competente in tema di ripristino della sicurezza in questi casi. e le georisorse) ha effettuato il sopralluogo e ha invitato il sindaco a recintare la zona, mettendo dei cartelli che attestano la pericolosità del luogo.

del 15 giugno 2010, firmata da vari colleghi di diversi Gruppi parlamentari. Si riferisce a un'ondata di multe anomale, dovute all'installazione di telecamere senza preavviso ai cittadini, presenti in varie zone di alcuni Comuni.

sollecito la risposta ad una serie di interrogazioni che riguardano la CONSOB. Ne ho presentate almeno 22

che gli atti di sindacato ispettivo sarebbero basati sul presupposto di plichi arrivati in forma anonima. in base a quale virtù taumaturgica - non so se fa l'indovino - questo signor Conti, presidente vicario, ancora oggi su «l'Unità» scrive una lettera dicendo

iniziative di un senatore della Repubblica: nessuno se lo può permettere, ne va della dignità del Senato. Non so se questo signor Vittorio Conti fa il presidente vicario o fa di professione l'indovino.

ho presentato esposti/denunce, tramite il Comando dei carabinieri del Senato, alle Procure delle Repubblica di Roma e di Milano per accertare se all'interno di questa CONSOB, di queste autorità pseudo-indipendenti, avvengano fatti

che hanno ridotto sul lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori e messo in mezzo alla strada le famiglie. Ringrazio per l'attenzione e auspico che il Governo, nella persona del Ministro dell'economia e delle finanze, venga a rispondere su fatti di una gravità estrema: non per l'indipendenza di queste

internazionale sull'AIDS. Il nostro Governo non ha deciso di partecipare con una rappresentanza governativa, ma soltanto diplomatica, e, cosa ancor più grave, non ha fatto sapere ai convenuti quali siano le sue intenzioni relativamente al conferimento delle due quote promesse, ma non mantenute, di finanziamento al fondo ONU su AIDS, malaria e tubercolosi. Si tratta di due *tranche* di 130 milioni di dollari promesse dal Governo Prodi e non mantenute dal Governo Berlusconi: il Governo Prodi, però, aveva soltanto incrementato quanto stabilito dal Governo Berlusconi nel 2001 al momento della creazione del fondo stesso. Ne va non soltanto della credibilità del nostro Governo nel consesso internazionale delle Nazioni Unite in materia di salute e di di aiuto alle popolazioni bisognose, in buona parte situate in Africa e in Asia centrale, ma anche del possibile boicottaggio di tutta una serie di programmi che avevano fatto conto su questi 260 milioni. Concludo il richiamo facendo anche notare che l'assenza del Governo italiano a quella Conferenza ha fatto sì che calasse la censura sui mezzi di comunicazione in Italia, perché non si è potuto vedere un solo servizio sulle reti radiotelevisive pubbliche relativamente alla riunione di Vienna. Ci sono ancora due giorni di tempo per rispondere.

di riduzione delle cosiddette spese per la rappresentanza politico-amministrativa nei Comuni, nello Stato, e così un ente come EUR Spa, che non è solo struttura romana ma ha anche carattere nazionale, proprietà al 90 per cento del Ministero dell'economia, nei mesi passati ha dato vita, nel silenzio generale e senza una procedura trasparente, alla creazione di tre nuove società. A noi pare che l'operazione sia francamente inammissibile e comunque incoerente. Vorremmo che il Governo desse una risposta circa la coerenza

della Commissione bilancio, la quale ha cercato di non esprimere un parere negativo. Invero, sull'unico articolo che riguarda i permessi di lavoro retribuiti (dieci all'anno) per le famiglie che perdono un familiare e non sanno dove sia finito, il Ministro dell'economia tiene in ostaggio la destra, la sinistra e il centro di questo Paese. Credo che qualsiasi funzionario, anche solo di buon cuore, del Ministero dell'economia che ha sotto gli occhi questa richiesta debba dare risposta alla 5a Commissione e permetterci di proseguire l'esame del

del collega. Il testo è stato presentato, spero che la Commissione bilancio possa avere al più presto la possibilità di esprimere il proprio parere. D'altra parte, ritengo ingiusto che un problema così importante e serio sia affrontato nel nostro Paese

(l'Italia è *market leader* a livello mondiale nella produzione di questi prodotti). Ebbene, queste aziende rischiano di fallire o di fuggire in altri Paesi

a quanto avvenuto negli altri Paesi europei, delle norme comunitarie, che evidentemente dà un potere assurdo e insensato ai timbri della burocrazia,